L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna. **Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni**

interministeriale MIUR-funzione pubblica), su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, sono dichiarate le equipollenze tra titoli di studio soltanto nei casi previsti dalla legge o dai bandi di concorso in conformità con la sentenza n. 3225/2005 del TAR Lazio e con la sentenza n. 830/1998 del Consiglio di Stato). Le proposte di equipollenza sono ad iniziativa delle università interessate e nel previgente ordinamento sono state dichiarate equipollenti numerose lauree rintracciabili, insieme ai riferimenti normativi, sul sito del Ministero. Per quanto riguarda le lauree specialistiche e magistrali, le equipollenze tra quelle del vecchio ordinamento non possono essere applicate ad esse per via transitiva in quanto le università hanno la possibilità di istituire numerosi corsi di studio afferenti ad una stessa classe ed aventi, tutti, lo stesso valore legale. Infatti, il decreto interministeriale del 9 luglio 2009 ha equiparato i diplomi di laurea del vecchio ordinamento con le classi delle lauree specialistiche e magistrali, ma l'equiparazione può essere attribuita, a seconda del percorso di studi seguito dallo studente, alternativamente ad una sola di esse; ai sensi dell'articolo 2 del suddetto decreto, l'università che ha conferito il diploma di laurea rilascerà, su richiesta dell'interessato, un certificato che attesti a quale singola classe è equiparato il titolo di studio posseduto. Come previsto dalla direttiva n. 3 del 2005 della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento funzione pubblica, le pubbliche amministrazioni, nella loro più ampia discrezionalità, nel prevedere i titoli richiesti per l'ammissione ai concorsi in relazione ai servizi ed alle funzioni che l'amministrazione stessa è chiamata a svolgere, sono obbligate al rispetto dei principi ordinari di valutazione delle equipollenze tra i titoli di studio secondo quanto previsto dalle norme legislative e dai decreti ministeriali. Tanto premesso, per quanto riguarda il concorso per commissari di Polizia di Stato, si ritiene che il Ministero dell'interno, nell'emanare il relativo bando, abbia operato in applicazione della suddetta direttiva.

mentre il Ministero dell'interno, nel bandire questo concorso per commissari di Polizia di Stato, avrebbe escluso i laureati in scienze della comunicazione

la legittima apprensione manifestata dal senatore Berselli in relazione alla notizia di stampa riguardante l'asserita sparizione dalla procura di Bologna di alcuni fascicoli di indagine, per quanto condivisibile, risulta essere assolutamente infondata. Mi pregio di comunicare, infatti, che la notizia della sparizione dei 2.321 fascicoli processuali, divulgata da quotidiani locali e nazionali, non trova riscontro nella realtà dei fatti ed è, piuttosto, il frutto di una fantasiosa ricostruzione giornalistica, tanto eclatante quanto inutile. Sia gli accertamenti compiuti *in loco* dal capo dell'ufficio, sia l'ispezione ministeriale del novembre 2008 - che pure, in prima battuta, aveva ipotizzato un'inattendibilità dei dati statistici per presunte irregolarità delle iscrizioni al Registro generale dei fascicoli di indagine - hanno definitivamente chiarito l'equivoco, spiegando i motivi dell'apparente disfunzione che tanto scalpore ha destato nei non addetti ai lavori. L'asserito mancato rinvenimento di numerosi fascicoli di indagine è dipeso, invero, dall'interpretazione non corretta della prassi gestionale in essere presso la procura bolognese e dalla conseguente errata individuazione del numero di fascicoli iscritti dal predetto ufficio giudiziario nel Registro generale. Intendo chiarire, infatti, che non di sparizione si è trattato, ma di semplice annotazione preventiva nei registri della procura dell'avvenuta definizione dei procedimenti di indagine, ancor prima dell'effettiva trasmissione al tribunale del fascicolo cartaceo. per esigenze organizzative dell'ufficio requirente bolognese, le annotazioni sono state anticipate all'atto dell'emissione del decreto di citazione in giudizio, quando il fascicolo non era stato ancora materialmente trasmesso al tribunale, perché in attesa del completamento degli adempimenti di segreteria. Nessuna sparizione di fascicoli, quindi, né - come riportato dalla stampa -armadi in cui gli stessi sarebbero stati rinvenuti, bensì semplici discrasie nella rilevazione numerica dei fascicoli pendenti, da cui non discendono profili disciplinari meritevoli di approfondimento, né condotte rilevanti ai sensi del decreto legislativo n. 109 del 2006. Faccio comunque presente che le autorità giudiziarie competenti, al fine di evitare futuri difetti di rilevazione statistica

una quota del gettito fiscale di competenza della Regione Lazio, nonché una parte delle quote del Fondo sanitario nazionale, di competenza della Regione Lazio, connesse all'attuazione degli obiettivi chiediamo di sapere se è possibile intervenire finanziariamente con anticipazioni nei confronti della Regione Lazio, tenendo conto che la situazione è particolare: c'è una forte esposizione debitoria ed è previsto un piano di rientro

possibilità di pagamento per le strutture convenzionate, per gli ospedali religiosi e per le tredicesime del personale dipendente. A queste domande, che abbiamo posto

Alla pagina 2 di tale nota, il ministro Sacconi scrive: «Relativamente alle somme riferite all'anno d'imposta 2007, di cui si chiedeva l'anticipazione, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato erogherà, a breve, 357 milioni di euro, sulla base del dato consuntivo». È stata data quindi una prima risposta affermativa per 357 milioni di euro. Vi è poi una seconda risposta, al punto 2),

del Governo se può confermare questo dato. A me risulta, in verità, che non tutto quello che il ministro Sacconi ha scritto il 3 dicembre alla Regione Lazio si è verificato, nel senso che

in questo curioso meccanismo, per il quale c'è un Patto di stabilità, un piano di rientro, un Commissario governativo, un'inadempienza - direi a questo punto

nel ripercorrere le vicende legate al dissesto dei conti sanitari della Regione Lazio, che hanno portato alla necessità di adottare il piano di rientro, chiedono di sapere se sia intenzione del Governo anticipare, prima della fine dell'esercizio 2009, una quota del gettito fiscale regionale, nonché una quota del Fondo sanitario nazionale. Al riguardo, si fa presente che l'erogazione delle spettanze residue a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, pari a circa 1.730 milioni di euro, è subordinata, ai sensi dell'ordinamento vigente, alla verifica positiva degli adempimenti previsti dal piano di rientro. Ove la Regione non adempia agli obblighi del piano, come è avvenuto per la Regione Lazio, sono sospese le erogazioni delle quote del maggior finanziamento del Servizio sanitario nazionale (quote premiali del finanziamento ordinario, fondo transitorio di accompagnamento dei piani di rientro e concorso statale ai ripiano dei disavanzi sanitari). L'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 189 del 2008, ha previsto la possibilità, con deliberazione del Consiglio dei ministri, di erogare in tutto o in parte le quote di finanziamento condizionate alla verifica positiva degli adempimenti in favore delle Regioni sottoposte ai piani di rientro e soggette a commissariamento per l'attuazione degli stessi. Tale possibilità è subordinata al verificarsi di due condizioni date dalla situazione di emergenza finanziaria nella Regione e dall'adozione, da parte del Commissario *ad acta* per l'attuazione del piano, di provvedimenti significativi in termini di effettiva e strutturale correzione degli andamenti di spesa sanitaria. Ai sensi del citato decreto-legge, le deliberazioni del Consiglio dei ministri che hanno autorizzato pagamenti in favore di Regioni sottoposte ai piani e commissariate, hanno fissato l'entità del pagamento in proporzione alla manovra correttiva effettivamente realizzata, rispetto alla manovra complessiva da realizzare. La Regione Lazio si è, peraltro, avvalsa di questa possibilità e a seguito dei risultati delle riunioni di verifica del 26 novembre 2008 e 1° aprile 2009, il Consiglio dei ministri, in data 28 novembre novembre 2008 e 22 maggio 2009, ha disposto in favore della Regione l'erogazione rispettivamente di 1.300 milioni di euro e di 828 milioni di euro. In particolare, la delibera del 22 maggio 2009 prevedeva anche la possibilità per la Regione di accedere all'erogazione di un ulteriore importo di 337 milioni di euro, subordinatamente alla verifica positiva da parte dei tavoli tecnici dei provvedimenti commissariali di modifica ed integrazione degli atti che presentavano criticità. Nella riunione di verifica tecnica tenutasi il 4 agosto 2009, relativamente alla possibilità di erogazione della predetta quota residua di 337 milioni i tavoli tecnici hanno valutato che non sussistevano i presupposti per procedere al pagamento in favore della Regione, ferma restando la sospensione dell'erogazione dei restanti 1.400 milioni di euro circa, in funzione della mancata completa realizzazione della manovra strutturale di contenimento dei costi prevista dal piano di rientro. Successivamente, il 10 novembre 2009, si è tenuta la riunione dei tavoli tecnici, nel corso della quale non sono emerse novità rispetto alla situazione riscontrata il 4 agosto e, pertanto, la riunione è stata aggiornata al 10 dicembre 2009. In ordine a quest'ultima riunione, gli esiti sono ancora in corso di formalizzazione. Con riferimento alle manovre fiscali regionali su IRAP e addizionale regionale all'IRPEF, per l'anno d'imposta 2007, a fronte dell'indicata somma da parte della Regione di 373 milioni di euro, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sta procedendo, come per tutte le Regioni interessate, al pagamento del saldo della manovra, pari a circa 357 milioni di euro sulla base del dato consuntivato dal competente Dipartimento delle finanze a novembre 2009. Per l'anno d'imposta 2008, si fa presente che la somma indicata dalla Regione in 936 milioni di euro è da rideterminarsi in circa 870 milioni di euro sulla base del dato stimato dal Dipartimento delle finanze. Rispetto a tale ultimo importo, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato: a) sta erogando alla Regione nel corso dell'anno 2009 tutte le quote affluite in tesoreria nel medesimo anno (parte dell'IRAP e l'intero gettito dell'addizionale regionale all'IRPEF) per un importo pari a circa 465 milioni di euro. Ciò in attuazione delle disposizioni recate dall'articolo del decreto-legge n. 112 del 2008, che prevedono, a decorrere dall'anno 2009, il trasferimento alle Regioni, nel mese successivo alla riscossione, di tutte le somme affluite sui conti di tesoreria a titolo di IRAP e di addizionale regionale all'IRPEF; b) sta procedendo ad anticipare a tutte le Regioni una quota del 60 per cento dell'acconto IRAP (affluito in tesoreria nell'anno 2008). Tale quota per la regione Lazio risulta pari a circa 243 milioni provvederà ad erogare a tutte le Regioni nel corso dell'anno 2010, in conseguenza della consuntivazione dei gettiti relativi all'anno d'imposta 2008, la restante quota dell'acconto IRAP, che per la regione Lazio è ad oggi stimabile in circa 162 milioni Per l'anno d'imposta 2009, si fa presente che la somma indicata dalla Regione in 911 milioni di euro è da rideterminarsi in circa 870 milioni di euro sulla base del dato stimato dal Dipartimento delle finanze. In ogni caso, tale ultimo importo affluisce solo in parte in tesoreria nell'anno 2009 (acconto IRAP, nel mese di dicembre), per un valore stimabile in circa 395 milioni di euro. È, peraltro, da segnalare che il gettito del mese di dicembre

circa 475 milioni di euro, affluirà in tesoreria nel corso dell'anno 2010 e, pertanto, allo stato risulta impropria la richiesta di erogazione da parte della Regione. Conclusivamente, con riferimento all'intero importo dei gettiti fiscali, pari a circa 2.220 milioni di euro secondo quanto riportato nella nota della Regione, da rideterminarsi in circa 2.100 milioni di euro sulla base delle più recenti stime del Dipartimento delle finanze, una quota pari a circa 1.460 milioni di euro è già stata erogata o verrà erogata entro il prossimo mese di gennaio (di cui circa 1.065 milioni di euro entro dicembre 2009). La restante parte, pari a circa 640 milioni di euro, sarà messa a disposizione della Regione nel corso dell'anno 2010, trattandosi per lo più di somme che debbono essere per l'appunto riscosse in tale anno. Si segnala, infine, che tutte le risorse in argomento sono finalizzate al settore sanitario. Qualora, invece, le stesse dovessero essere utilizzate dalla Regione sul piano della cassa per altre finalità, si aggraverebbero ulteriormente le tensioni finanziarie nel settore. ultimo, per quanto attiene le erogazioni, in corso di predisposizione, delle quote di manovra fiscale regionale indicate nella misura complessiva di circa 600 milioni di euro, si soggiunge che queste avverranno nella settimana compresa fra il 15 ed il 23 dicembre 2009.

cui saranno erogate le somme spettanti alla Regione. Questa è una buona notizia perché in questa sede, cioè nell'Aula del Senato, un'affermazione di questo genere ha un valore maggiore che non una lettera del Ministro.

(spesso i quesiti logici sono più duri di quelli politici): come fanno i cittadini del Lazio ad essere impegnati a pagare sovrattasse per l'IRAP e per l'IRPEF, che vengono poi

perché è ben buffo un ordinamento nel quale io nomino il commissario, il commissario da me nominato non raggiunge risultati e tu paghi. Non credo sia un problema di destra o di sinistra: è che qualche volta, nel fare le leggi, dovremmo riflettere meglio. Credo sia un impegno *bipartisan*, se così possiamo dire, per questo lavoro che dobbiamo fare ora che in finanziaria tornano le regole del Patto della salute. Le sarei davvero grato, signor Sottosegretario, se considerasse questo aspetto critico della normativa che abbiamo fin qui sviluppato, perché forse il Governo, in sede di Conferenza Stato-Regioni, dovrebbe pur sollevare la questione e riflettere insieme alle Regioni sulle soluzioni da proporre al Parlamento.